il provvedimento al nostro esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, offre un quadro di riferimento organico agli investitori, capace di stimolare l'intensificazione dei rapporti economici tra Italia e Malawi. Esso rappresenta per gli investitori italiani una prospettiva di applicazione delle migliori condizioni, anche fiscali, per i loro investimenti e mira a fornire la garanzia della possibilità di libero trasferimento degli utili e dei capitali e dell'applicazione di criteri imparziali in caso di controversie. Il Malawi è da considerarsi un Paese interessante soprattutto per le prospettive di sviluppo: tuttora, infatti, il reddito medio *pro capite* della popolazione è molto basso, ma negli ultimi anni, pur in presenza della grave crisi finanziaria internazionale, il tasso di crescita del Paese si è mantenuto sempre al di sopra del 4 per L'Accordo, che si compone di 16 articoli, reca una norma iniziale relativa alle definizioni, tra le quali appare significativa quella relativa all'«investimento», che ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del Paese contraente. In base all'articolo 2, l'applicazione dell'Accordo riguarda in via esclusiva gli investimenti nel territorio di una parte contraente, effettuati da cittadini o società dell'altra parte, approvati dall'autorità competente designata dalla parte nel cui territorio avviene l'investimento, alle condizioni da questa fissate. L'Accordo si applicherà anche agli investimenti precedenti l'entrata in vigore di esso, e indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche tra le parti. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle parti si impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati, nonché la libertà di soggiornare - con i loro familiari - nel territorio dell'altra parte per il periodo necessario, durante il quale potranno liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità. Le parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di Paesi terzi, con l'eccezione dei benefici concessi da una delle parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a livello regionale a unioni economiche o a zone di libero scambio. La clausola della Nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari. La protezione degli investimenti è assicurata inoltre dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Ognuna delle due parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati: anche a tali trasferimenti sarà applicabile la clausola della Nazione più favorita. In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra parte la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato. Per le controversie di cui all'articolo 11, in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali della parte contraente avente giurisdizione territoriale, da un lato, e l'arbitrato internazionale - quale previsto dai regolamenti della Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale - dall'altro. Le controversie fra parti, disciplinate dall'articolo 12, prevedono invece il ricorso eventuale a un tribunale arbitrale *ad hoc*. L'articolo 14 permette alle parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle parti contraenti, nonché di ricevere un indennizzo in caso di inottemperanza di una delle parti a tali previsioni. La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza. L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento.

Signor Presidente, inizio con una questione relativa all'organizzazione dei nostri lavori: fino a ieri pomeriggio non erano chiari i termini per la presentazione di documenti che potessero accompagnare

in molte occasioni - ne parleremo in seguito relativamente alla Bielorussia - si firmano accordi bilaterali con Paesi che non necessariamente eccellono in due campi fondamentali per l'impegno internazionale del nostro Paese:

forse va collocato in un contesto in cui in Africa c'era ancora la speranza di poter vedere investimenti occidentali

dei problemi, da aggiungere alle persecuzioni per identità di genere o orientamento sessuale, che sono stati sulle pagine di tutti i giornali all'inizio dell'anno. Un Malawi che nella classifica di *Transparency International*, resa pubblica un paio di giorni fa, non svetta tra i Paesi con

non solo non ha una ambasciata in Malawi, ma l'ambasciata competente per il Malawi, che si trova nello Zambia, a Lusaka, da 11 mesi non ha un ambasciatore. Purtroppo, salvo che non sia in arrivo, non c'è un rappresentante della Farnesina in Aula nel momento in cui si ratifica questo Accordo. È bene però che si sappia che, se si ritiene di dover avere un rapporto bilaterale talmente forte da dover andare a ratificare un trattato, allo stesso tempo, conoscendo la controparte di questo Accordo, occorre, se non altro, essere presenti sul territorio per verificare quotidianamente che esso venga applicato. non dico di aprire una ambasciata in Malawi, fatto che sicuramente, visti i tagli che caratterizzano il Ministero degli affari esteri, è impossibile, ma se non altro dotare quella di Lusaka di un ambasciatore che - ripeto - manca da 11 mesi. La cosa che sarebbe stata anche utile acquisire agli atti è il volume di affari reciproco. Dubito che ci sia un imprenditore del Malawi che abbia speso una lira che non sia in *shopping* in Italia e che quindi abbia voluto investire nel nostro Paese. Dubito allo stesso tempo che ci sia tutta questa necessità di correre in Malawi ad investire in un contesto - ripeto - in cui il privato sicuramente ha altri tipi di opportunità di essere presente nel settore economico, mentre il pubblico negli ultimi dieci anni si è ritirato, arrivando ad essere presente per lo zero per cento dei progetti di cooperazione bilaterale con quella parte dell'Africa. la raccomandazione, che avrei voluto fare per iscritto ma che faccio oralmente, è che, se non altro, essendoci un'ambasciata nello Zambia, si passi a brevissimo termine alla nomina dell'ambasciatore. Tale ambasciata oggi è retta da un efficiente ed efficace incaricato d'affari - che, peraltro, è stato fondamentale in una missione che due settimane fa, assieme alla deputata radicale, Elisabetta Zamparutti, abbiamo fatto nello Zambia per perorare la causa della abolizione della pena di morte - il quale si trova ad avere a che fare non con i suoi pari, ma con ambasciatori di rango, che chiaramente vengono presi in considerazione magari prima del nostro incaricato di affari, quando ci sono dei rapporti con il Governo locale.

invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente

ai relativi oneri, di carattere eventuale e connessi al verificarsi degli eventi indicati dalla norma (conflitto armato, stato d'emergenza, conflitti civili), si farà fronte con autonomi provvedimenti connessi agli specifici eventi».

vorrei aggiungere alcune considerazioni. Innanzitutto, concordo con molte delle osservazioni fatte in sede di discussione generale dal collega Perduca, che fa bene a porre delle problematiche, però va anche ricordato che

assaliti da problematicità e criticità. L'aspetto positivo di questo provvedimento è proprio il fatto che esso mira, quantomeno sulla carta, ad incentivare lo sviluppo nei Paesi più poveri con

poiché le buone intenzioni rispetto alle politiche di sviluppo dei Paesi poveri non possono che essere apprezzate.

tra qualche giorno nella discussione sulla manovra finanziaria, come quella di una riduzione veramente impressionante dell'aiuto italiano allo sviluppo e delle risorse destinate alla cooperazione, in particolare

non ci possiamo considerare con la coscienza a posto semplicemente ratificando questo Accordo, poiché ci sono problemi molto grandi che riguardano le nostre scelte e che dovremo affrontare. Ricordo solo che il Regno Unito il giorno stesso in cui ha deciso un'operazione di taglio di quasi mezzo milione di posti di lavoro, cioè un'operazione gigantesca

esattamente nella direzione opposta rispetto a quella di un Paese che sa quale sia il suo ruolo nel mondo.

Occorre evidenziare in questo caso che si tratta di interventi non invasivi, cioè di interventi che hanno anche lo scopo, non dichiarato ma concretamente realizzabile, di far progredire quei Paesi in cui, come diceva il collega Perduca, i diritti umani, la democrazia e la libertà religiosa sono ancora veramente temi molto lontani dall'essere acquisiti.

a quei Paesi che debbono ancora avviare un processo di democratizzazione interna. Vorrei sottolineare, in ogni caso, che in particolare l'Accordo con questo Paese

condizioni la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale,

Sappiamo, ahimè, che, per prassi, si pongono all'ordine del giorno le ratifiche dei trattati come riempitivo, e spesso si tratta di trattati molto importanti, non soltanto nel merito, ma anche nella selezione del partner. La Bielorussia è sicuramente uno di questi casi di scuola. La Bielorussia, assieme alla Russia e alla Libia, è stata eletta dal Presidente del Consiglio dei ministri come partner principale e strategico nelle relazioni internazionali che il nostro Governo intrattiene, sorpassando, che so, gli Stati Uniti, la Germania e la Turchia, per citare tre Paesi con i quali invece il volume di affari è fondamentale per lo sviluppo della nostra economia nel settore delle esportazioni. La Bielorussia - credo occorra a questo punto ricordarlo all'Aula - è un Paese che dal 1996 ha deciso di abolire la possibilità di limitare la rielezione del Presidente (magari, diciamo così, in questo amore spassionato nei confronti di Lukashenko, il Presidente del Consiglio proietta alcuni dei propri desideri) l'aver tolto i limiti alla rielezione ha fatto sì che, da oltre vent'anni, ci sia lo stesso Presidente in quel Paese. Nel corso delle ultime elezioni parlamentari, tenutesi nel settembre del 2008 in Bielorussia, non è stato eletto - pensate un po' - nessun rappresentante dell'opposizione e l'intero processo elettorale è stato considerato dall'OSCE non trasparente né, quindi, legittimo. il prossimo 19 dicembre si terranno le prossime Elezioni Presidenziali e che durante la campagna elettorale, presumibilmente, non verrà garantita la libertà di espressione ai candidati dell'opposizione e saranno caratterizzate da massici brogli elettorali; la Bielorussia è l'unico dei Paesi Europei e dell'ex-Unione Sovietica che pratica ancora la pena di morte, per 14 reati. Non si hanno dati precisi in quanto tutte le notizie a riguardo sono soggette al segreto di stato,

a causa del mantenimento della pena di morte, è l'unico paese della regione escluso dal Consiglio d'europa; sappiamo però che è in corso un dibattito, almeno a parole, in quel Paese per arrivare all'abolizione della pena di morte e sappiamo anche che l'Italia, grazie alle iniziative dei radicali, dal 1992-1993 è uno dei Paesi capofila della promozione dell'abolizione della pena di morte e di una risoluzione alle Nazioni Unite che chieda la sospensione, una moratoria, di tutte le esecuzioni capitali nel mondo.

una condizione che prepara al dialogo su altri temi) e di richiedere alcune decisioni a livello nazionale. Ma tutte le volte che si va alla corte di Lukashenko di tutto si parla tranne che, per esempio, della moratoria della pena di morte o dell'unione della Bielorussia al fronte di coloro che alle Nazioni Unite si battono contro la pena di morte. Queste denunce provengono sia dalle organizzazioni non governative attive in in clandestinità in Bielorussia, che da quelle internazionali che seguono le violazioni dei diritti umani, ma anche dal Dipartimento di Stato americano (non propriamente un'organizzazione dedita alla promozione e protezione dei diritti umani in maniera in maniera *super partes*). Nel rapporto sui diritti umani del 2009, pubblicato l'11 marzo di quest'anno, vengono analizzate nel dettaglio le carenze democratiche riscontrate in Bielorussia e si riporta una lunga lista di problemi, che crediamo debbano essere posti all'attenzione del nostro Parlamento. Se dovessimo limitarci a ciò che è di dominio politico, certamente è impossibile fare, dal punto di vista della partecipazione elettorale, opposizione al regime di Lukashenko, perché si sistematicamente arrestati con detenzioni arbitrarie per motivi politici. Il caso più esemplare è quello di Alexander Kozulin, già candidato alle elezioni presidenziali nel 2006 e privato della libertà per oltre due anni.

a tenere un approccio molto morbido nei confronti di Lukashenko, il quale, ricordiamolo, è il presidente di un Paese attraverso il quale passa buona parte del gas e del petrolio proveniente dalla Russia e destinato ai mercati europei. Altre organizzazioni, come *Reporters sans frontières* riferiscono che la Bielorussia occupa il 154° posto, su 178 Paesi esaminati, dal punto di vista della libertà di stampa, che Internet ormai è stata messa sotto il controllo del Governo: un Governo che ha mantenuto in piedi l'impalcatura del KGB di eredità sovietica.

si impegna il Governo a «chiedere al Consiglio dell'Unione europea di rivalutare la propria linea morbida nei confronti del Governo di Minsk e di vincolare il proseguimento del dialogo con le autorità bielorusse all'immediata liberazione dei due prigionieri politici Mikalay Autukhovich e Uladzimir Asipenka, all'introduzione di una moratoria sulla pena di morte e alla tenuta di elezioni libere e democratiche il prossimo 19 dicembre». poiché in passato non soltanto sono stati messi in carcere leader politici, non soltanto è stata pressoché abolita la libertà di espressione a mezzo stampa, ma è stata anche chiusa una delle poche università indipendenti che operava in quel Paese, si chiede all'Italia di «unirsi ai 14 Governi europei che sostengono finanziariamente l'Università per gli studi umanistici, chiusa dalle autorità bielorusse nel 2004 e che ora opera in esilio a a Vilnius accogliendo ogni anno centinaia di studenti bielorussi, tra cui coloro che per motivi politici vengono espulsi dagli atenei del Paese e privati del diritto allo studio». Oggi ci accingiamo a ratificare

allora che il Governo - magari limando alcune parti del dispositivo, se si ritiene che sia troppo stringente

del diritto internazionale (che comunque negli ultimi 40 anni sono stati codificati in strumenti dei diritti umani internazionali, che l'Italia ha puntualmente ratificato, anche se talvolta stenta nell'applicarli quotidianamente), ma di vite umane, che qui sono alla mercé di uno Stato non democratico.

quando si parla della Bielorussia, è giusto che sia ogni volta ricordato tratta non solo di un Paese che è l'unico dei 47 membri del Consiglio d'Europa che continua a emanare condanne a morte e ad eseguire sentenze capitali,

scegliamo la strada del dialogo e del confronto, perché può permettere di cambiare la situazione e di aprire una fase nuova che riporti quel Paese nell'ambito della comunità democratica,

sarebbe un orientamento sbagliato, che l'apertura del dialogo comporti la rimozione, l'impegno a tacere, a mettere sotto il tappeto, a non guardare contraddizioni così vistose.

punto provo a proporre una riformulazione: si potrebbe impegnare il Governo a chiedere al Consiglio dell'Unione europea che nel dialogo con il Governo di Minsk sia posta con forza la richiesta della liberazione dei due prigionieri politici, dell'introduzione di una moratoria sulla pena di morte e della tenuta di elezioni libere e democratiche.

segnalo che anche in Italia vi sono state iniziative di accoglimento di studenti bielorussi espulsi per ragioni politiche dalle università bielorusse (ad esempio, ciò è avvenuto nella città di Milano). Ritengo, pertanto, che anche questo secondo richiamo, almeno come invito al Governo a considerare tale possibilità, debba essere preso in esame.

vorrei ribadire in questa sede il serio impegno del Governo italiano per il rispetto dei diritti umani, nonché il convinto appoggio che il nostro Governo ha dato all'Alto rappresentante dell'Unione europea

Grazie passiamo al successivo

e non solo per tutto quello che ha significato quella parte dell'Europa nel passato, ma anche e soprattutto per il fatto che la Slovenia è ormai parte integrante dell'Unione europea

una pagina buia e oscura che ha conosciuto la storia europea negli anni passati. Per tornare al significato del provvedimento, nell'ottobre 1980 i Governi italiano e jugoslavo firmarono a Nuova Gorizia un accordo per la manutenzione del confine, onde assicurare l'integrità e la visibilità dei cippi che segnano la frontiera tra i due Stati, fissata dal Trattato di pace di Parigi del 1947 e dal Trattato di Osimo del 1975. Nel 1991, con la nascita della Repubblica di Slovenia, subentrata alla Jugoslavia come parte contraente dell'Accordo, le problematiche di confine conseguenti al nuovo quadro politico sono state riviste e sono state inoltre prese in considerazione le possibilità messe a disposizione dall'evoluzione tecnologica. Ciò ha indotto il Governo di Lubiana a chiedere la conclusione di una convenzione, che è stata preceduta, a partire dal 1998, da una nuova misurazione generale dell'intero confine di Stato con metodologia satellitare. Il risultato delle operazioni di rilevamento, concluse nel 2004, è stato documentato dalla Commissione mista per la manutenzione del confine di Stato attraverso specifici documenti tecnici che costituiscono parte integrante della nuova Convenzione. L'Accordo in questione mira altresì a regolamentare in modo più puntuale i lavori di manutenzione e di visibilità dei termini e del tracciato del confine secondo le rispettive competenze ed a garantire agli incaricati dei lavori l'attraversamento della linea di confine e gli eventuali indennizzi a terzi che ne potrebbero derivare. La Convenzione definisce, inoltre, le limitazioni di eventuali costruzioni in prossimità del confine ed istituisce una Commissione mista con lo scopo di dirigere e regolamentare tutti i lavori e un gruppo misto di esperti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine. Ai membri della Commissione mista ed alle persone incaricate dei lavori di manutenzione è assicurata l'immunità personale e l'inviolabilità dei carteggi al seguito. Il disegno di legge di conversione contiene, oltre alla consueta norma di autorizzazione alla ratifica ed all'ordine di esecuzione, una disposizione sulla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo. L'onere complessivo ammonta a 32.705 euro per l'anno 2010, a 19.000 euro per l'anno 2011 ed a 32.705 euro annui a decorrere dall'anno 2012. Nel corso della prima lettura è stato approvato un emendamento che specifica le modalità di monitoraggio degli oneri. Come vede, Presidente, non è consuetudine dei relatori della 3a Commissione entrare troppo nel merito dei testi e leggerli per intero.

onorevoli colleghi, è senza dubbio positivo fissare, con maggiore chiarezza giuridica, il tracciato del confine di Stato fra Italia e Slovenia nonché responsabilità e competenze per la manutenzione dello stesso, di modo da rispettare quanto dal Trattato di pace di Parigi del 1947 e dal Trattato di Osimo del 1975. Il confine con la Slovenia, tuttavia, non ha solo un significato geografico o amministrativo, ma possiede un forte valore politico e culturale: dal 2004, infatti, la frontiera è stata aperta e l'estremo limite dell'Europa occidentale, separato dalla cortina di ferro rispetto ai Paesi del Patto di Varsavia, è caduto. Quel confine, per tanti anni, è stato un confine ideologico fra capitalismo e comunismo, fra economia di mercato ed economia del socialismo reale, e sul quel confine, o meglio in nome di quel confine e della paura di una sua modifica per la supremazia di una visione del mondo sull'altra, si sono combattute tante guerre e tanto sangue è stato sparso, dal Vietnam alla Corea alle guerre "per procura" in Africa. Esprimo, pertanto, il voto favorevole dell'Italia dei Valori al Trattato internazionale fra l'Italia e la Repubblica di Slovenia, subentrata alla Jugoslavia come parte contraente dell'Accordo nel 1991, auspicando che oggi, anche in vista dell'ingresso di molti Paesi ex jugoslavi in Europa, prima fra tutti la Croazia, il portato politico e valoriale associato al confine sia capovolto per diventare una potenziale risorsa di scambio economico e culturale con i Paesi dell'area balcanica. Bruxelles ormai da anni, dalla conclusione dei due conflitti nell'area della ex Jugoslavia, sta guardando ad Est e la politica di integrazione messa in atto è volta proprio alla determinazione di un processo di stabilizzazione, di pace e di prosperità. A tutto questo, le relazioni italo-slovene possono dare un contributo importante, che si fissa innanzitutto con l'atto in discussione oggi. Invito altresì il Governo a prendere la discussione di oggi come spunto per chiudere le tensioni per chiudere le tensioni e gli aspetti non risolti che riguardano le ferite non ancora rimarginate di quei conflitti intorno alla cortina di ferro. C'è il Trattato di Osimo, ci sono i beni dei nostri italiani che si sono dovuti allontanare da quelle terre e per i quali noi dell'Italia dei Valori, ma anche altre forze politiche del Parlamento, abbiamo presentato proposte di legge tese a risolvere una volta per tutte questo annoso e irrisolto problema nazionale di dignità dei nostri cittadini. Il Governo deve agire, così come per gli espatriati libici, per ridare loro la dignità e l'uguaglianza come cittadini italiani a pieno titolo. È tempo di dare le risposte che tanti connazionali ancora oggi attendono.

di fatto questa Convenzione rispetto ad altre sembra avere un impatto non molto impegnativo, ma certamente, una volta approvata, riteniamo che essa chiuda un percorso lungo di rapporti e convenzioni tra il nostro Paese e la ex Jugoslavia.

Le popolazioni, sia da una parte che dall'altra, sono sempre le stesse, ma le esperienze e i confronti che in questi anni si sono verificati, quando quel confine veniva chiamato cortina di ferro, si sono determinate in modo molto preciso ed hanno lasciato purtroppo segni ancora profondi.

Di questo contenuto voglio sottolineare semplicemente quella parte che va a gestire, a cavallo del confine, i rapporti e i passaggi delle popolazioni e degli interessati, che dovrebbe agevolare una buona soluzione dei problemi ed una definitiva normalizzazione dei rapporti. È infatti opportuno che in futuro questa Convenzione sia la base giuridica e politica per andare oltre le difficoltà che si sono determinate in questi anni e superare in modo definitivo Se pensiamo che l'Europa si è allargata ed è arrivata a 27 Paesi, e si è allargata soprattutto verso Est, e che questo confine è diventato comunque un centro più che un confine rispetto all'allargamento ad Est, diventa fondamentale che si chiudano quelle tensioni, si chiariscano le incomprensioni che ancora persistono e si arrivi ad una situazione di pace e di collaborazione Non c'è più la Jugoslavia: c'è la Slovenia e, vicino, c'è la Croazia, che sta aspettando da tempo di entrare a far parte dell'Unione europea. Dobbiamo quindi fare attenzione alle tensioni che ancora esistono tra questi Paesi. Ritengo che il confine di Stato tra l'Italia e la Slovenia possa diventare veramente un confine aperto anche grazie a questa Convenzione: un confine ricco di proposte per migliorare il rapporto tra questi popoli guardando soprattutto ad Est. Pertanto, le motivazioni di fondo che dovranno muovere le future azioni anche del nostro Governo sono tutte all'interno di questa Convenzione, per farla diventare soprattutto un contenuto di proposta, una Convenzione che guardi ancora più lontano del momento contingente. Le preoccupazioni del passato devono diventare speranze e prospettive per il futuro. Per queste ragioni, riteniamo di esprimere in maniera convinta un voto favorevole alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. Art.

che è importante anche rispetto allo scenario futuro dell'area del Sud Est europeo. A nome del Gruppo Partito Democratico dichiaro il nostro convinto appoggio alla ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, già approvata dalla Camera. Si tratta di un atto formale con contenuti di carattere tecnico, che però racchiude in sé un valore politico. Mi permetto inoltre di svolgere alcune considerazioni rispetto ai rapporti di collaborazione tra i due Stati ed alle relazioni tra l'Italia e gli altri Paesi dell'ex Jugoslavia. Ne parlo perché sono convinta si tratti di un'area strategica, soprattutto nella prospettiva dell'ulteriore allargamento dell'Unione europea in un processo di stabilizzazione e di pace. Tornando alla Convenzione, vorrei ricordare alcuni avvenimenti che hanno radicalmente cambiato lo scenario del cosiddetto confine orientale. Esso è stato tracciato prima dal *Memorandum* di Londra e poi in maniera definitiva

è stato di fatto recepito anche il tracciato del confine. Stiamo parlando di un confine a lungo conteso, non solo dopo la fine della guerra, ma molto prima. Nel Novecento l'area del Nord Est Adriatico è stata teatro di gravi tensioni, di sofferenza e dolore; nel dopoguerra quel confine è stato segnato dalla guerra fredda ed ha rappresentato la divisione tra due sistemi sociali e politici diversi e contrapposti. La cortina di ferro, come l'ha chiamata Churchill, ha per lungo tempo contrassegnato negativamente la vita in quel territorio etnicamente plurale. Ma oggi abbiamo davanti a noi un nuovo scenario, in cui il confine ha un carattere puramente amministrativo: con l'entrata della Slovenia, nell'Unione europea il 1° maggio 2004, e poi nell'area Schengen il 21 dicembre 2007, si sono di fatto dissolte le barriere fisiche tra i due Paesi. È stato così definitivamente chiuso un periodo storico. Oggi tale confine è solamente una linea di demarcazione, attraverso la quale c'è la libera circolazione di beni e persone. È necessario cogliere le opportunità di sviluppo che offre quest'area, cercando di cancellare gli steccati che sono ancora rimasti nella coscienza delle persone, che sono di carattere psicologico, culturale, sociale e linguistico. Le differenze, i pregiudizi ed i sospetti vanno superati attraverso la conoscenza reciproca e la collaborazione, in particolare quella transfrontaliera. Come Partito Democratico stiamo chiedendo anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia un impegno maggiore in questa direzione. La Slovenia è oggi un Paese dinamico, membro affidabile dell'Unione europea, che ha anche presieduto con competenza e responsabilità; la lingua slovena è una delle lingue ufficiali dell'Unione. Recentemente, con l'approvazione dell'arbitrato con un *referendum,* ha fatto un passo decisivo sulla strada dell'entrata della Croazia nella Comunità europea. Per quanto riguarda l'Italia e la Slovenia, molto è stato fatto negli ultimi anni per migliorare i rapporti, ma si può fare di più, da ambedue le parti, perseguendo insieme obiettivi di più ampio respiro. Va ricordato che le principali questioni storiche tra i due Paesi sono state chiuse. In questo clima di amicizia si riuscirà a trovare la condivisione anche rispetto alle nuove sfide, dalle infrastrutture alle sinergie portuali, dalla politica energetica all'utilizzo dei fondi europei. A questo proposito, non posso non ricordare in quest'Aula il grande evento svoltosi a luglio di quest'anno a Trieste, e cioè il Concerto dell'amicizia, con la presenza dei tre Capi di Stato, italiano, sloveno e croato. In quella occasione, i tre Presidenti hanno visitato insieme due luoghi che testimoniano le tragiche vicende storiche di quelle terre: il Narodni dom, centro economico e culturale degli sloveni, bruciato nel 1920 dalla barbarie fascista, e la lapide a testimonianza del tragico esodo dall'Istria e dalla Dalmazia. Si è trattato di un atto di riconciliazione, di un atto simbolico che testimonia la volontà di guardare al futuro con speranza ed ottimismo, C'è la comune consapevolezza che quell'area, da periferia marginale, può diventare un'area competitiva e centrale dell'Europa e dare così alle nuove generazioni prospettive di crescita. Accenno brevemente ad un tema che assume un ruolo importante nelle relazioni tra i due Paesi e cioè quello delle minoranze, la slovena in Italia e la italiana in Slovenia: esse sono state, e saranno ancora di più nel prossimo futuro, un collante insostituibile in questi rapporti. È necessario, comunque, dare piena attuazione alle leggi vigenti e dimostrare la necessaria sensibilità nell'affrontare le diverse politiche riferite alle minoranze. In questo contesto, alcuni giorni fa, il presidente sloveno Danilo Türk ha incontrato a Pirano i rappresentanti della comunità italiana. È stato un incontro cordiale e significativo, in cui il Presidente ha ribadito la necessità di un maggiore impegno per le scuole italiane e la valorizzazione della lingua, dichiarando che la minoranza italiana sta dando un contributo importante allo sviluppo culturale complessivo della Slovenia. Auspico, perciò, una maggiore attenzione del Governo italiano rispetto all'attuazione della legge n. 38 del 2001, che dopo 10 anni è solo parzialmente applicata, ed in particolare rispetto al finanziamento delle attività culturali. culturali. Tralascio la questione dell'area del Sud Est degli ex Paesi iugoslavi, in cui i nostri due Stati, insieme, potrebbero fare molto di più, anche perché si tratta

rispetto a tale Convenzione, auspicando che essa possa essere approvata con il consenso di tutti i Gruppi, a dimostrazione che le cose sono davvero cambiate

Presidente, ho poco da aggiungere, dopo tutto quello che è stato detto. Si tratta di un provvedimento tecnico e, non per nulla, è stata istituita una Commissione mista con lo scopo di dirimere e regolamentare tutti i problemi tecnici che si pongono in questo quadro. Naturalmente, non ci siamo nascosti e abbiamo tutti

coloro i quali lo hanno sottolineato - per fortuna e finalmente si chiude una delle ultime pagine della storia del passato.

Richiamo e condivido quanto dichiarato in questo momento dal senatore Bettamio, a nome e per conto del Gruppo PdL, sugli aspetti tecnici del provvedimento ma, soprattutto, sull'armonizzazione, che ancora deve avvenire appieno,

della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004***

Il disegno di legge in esame tratta il negoziato tra la nostra Repubblica e quella di Azerbaigian, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmato il 21 luglio 2004. Innanzitutto bisogna premettere che, assieme a Georgia ed Armenia, l'Azerbaigian occupa quella zona che si trova fra Turchia, Iran e Russia, da cui il 18 ottobre 1991 si dichiarò indipendente. Questo Accordo viene applicato alle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti e si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio, tenuto conto della vigenza di imposte patrimoniali nel sistema fiscale Nello specifico si tratta di una Convenzione, simile agli altri Trattati per evitare le doppie imposizioni stipulati dall'Italia, basata sul modello OCSE di Convenzione, da cui si differenzia solo in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali italiano e azero. Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione in oggetto non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario. Concludo che è necessario approvare un Accordo per evitare le doppie imposizioni, disciplinando cosi gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e l'Azerbaigian, un Paese ricco anche di riserve minerali, tra cui gas naturale e petrolio, e riserve che possono essere impiegate nella metallurgia, nell'edilizia e nell'industria farmaceutica. Pertanto ritengo necessario approvare il disegno di legge in esame. **Testo

Siamo i terzi a livello di esportazioni (dico: purtroppo) verso il Paese e primi a livello di importazioni. Questo dovrebbe

occorre incrementare maggiormente la nostra presenza. Ce lo chiede anche il Governo azero. Si potrebbe intensificare questo settore, e le nostre imprese ne trarrebbero forti guadagni. Per tale ragione, occorre intervenire e non sottovalutare questa fase di espansione

Presidente, ringrazio il relatore per la puntuale esposizione. Concordo con l'intervento fatto in questo momento sull'importanza della ratifica, che si inserisce nel quadro della strategia bilaterale verso i Paesi del partenariato orientale dell'Unione europea, iniziativa tramite la quale il Ministero degli affari esteri mira, in parallelo con il progetto comunitario del partenariato orientale, a rafforzare i propri rapporti bilaterali con i Paesi coinvolti coinvolti (Bielorussia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia e, appunto, Azerbaigian) con un approccio inclusivo e multisettoriale a sostegno della cooperazione regionale, anche eventualmente mettendo a frutto gli strumenti offerti dall'Unione europea.

il sottosegretario Scotti, per aver capito e intuito tutte le potenzialità che questo Paese può dare alle imprese italiane.

l'interessante potenzialità che questo Paese ha sotto il profilo economico con il nostro. Importante può essere lo sviluppo, un incremento di investimenti del nostro Paese in Azerbaigian, sperando che non vi sia una delocalizzazione. L'invito, il vero obiettivo non è quello di trasferire le attività produttive collocate nel nostro territorio in Paesi Ovviamente la vera *ratio* è cercare di incrementare, sì, le attività economiche con i vari Paesi, ma ovviamente non necessariamente andando ad incentivare la delocalizzazione che, per come la penso io, è invece un problema e non qualcosa di positivo per quanto ci riguarda. Si tratta di una Convenzione simile a tutti gli altri trattati per evitare doppie imposizioni. Si differenzia solo in alcuni aspetti derivanti appunto dalla particolarità dei sistemi fiscali italiano e azero. azero. Quindi, ribadisco il voto favorevole della Lega Nord e consegno l'intervento

Il provvedimento in esame ha come oggetto la Convenzione tra Italia e Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali ed il relativo Protocollo.

sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al modello OCSE, tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria. L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia, la riforma del 1997 ha portato all'abolizione dell'ILOR e all'introduzione dell'IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari. La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana (articolo 2, paragrafo 3, lettera riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che ora deve intendersi sostituita dall'IRES, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive. In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione. Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interesse dei due *partner* negoziali. Per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte,

Va peraltro rilevato che dell'aliquota del 5 per cento non possono beneficiare le cosiddette *non resident-owned investment corporations* le quali sono entità di diritto canadese che possono, all'occorrenza, essere utilizzate (ad esempio, nella forma di una società *holding* canadese) in modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possieda l'intero pacchetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Canada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rimborsi d'imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una *non resident-owned* *investment corporation* sarebbe pari alla ritenuta alla fonte prevista L'esclusione in questione è, pertanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresì gli investimenti diretti. Nel contesto dell'articolo è stata definita, altresì, la disciplina della cosiddetta *branch tax* (articolo 10, paragrafo 6). Tale imposta - in aggiunta alla normale imposta sul reddito - è generalmente applicata sul reddito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere che svolgono attività di compravendita immobiliare in Canada mediante una stabile organizzazione, con l'aliquota del 25 per cento (o inferiore, se prevista in base a una convenzione contro le doppie imposizioni). In tema di *capital gains* (articolo 13), è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi) che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato. Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un *tax deferral*, vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi. Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata ed in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni. La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa, in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. Si attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione. Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione sono stati condivisi ì principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi stipulati dal nostro Paese. Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto il metodo di imputazione ordinaria. Poiché la presente Convenzione, allorché entrerà in vigore, sostituirà la vigente, è stata prevista anche una clausola di cessazione degli effetti, con una particolarità: se le disposizioni della cessanda Convenzione dovessero consentire trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all'ultimo giorno dell'anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni). In conclusione, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, data l'impossibilità di una quantificazione degli oneri sulle questioni rilevate e nel presupposto della sostanziale irrilevanza degli effetti di gettito, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

infatti inutile essere troppo ripetitivi, vista l'ottima relazione del senatore Giordano: una relazione chiara e completa.

non sottolineare come anche un provvedimento tecnico possa servire e contribuire utilmente a ricreare un clima di reciproca conoscenza e di apertura nei confronti di un Paese che oggettivamente, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, era tra quelli rimasti più indietro nei rapporti con l'Europa e con il mondo occidentale. Indubbiamente, rimangono una serie di perplessità

perché aprire un dibattito sulle premesse implicherebbe un'analisi attenta della situazione, delle cose che non vanno e di quelle che si possono e si devono fare.

la tenuta di elezioni libere e democratiche il 19 dicembre». Per quanto riguarda l'ultimo capoverso (pregando di soprassedere

chiusa dalle autorità bielorusse nel 2004 e ora operante a Vilnius, accogliendo ogni anno centinaia di studenti bielorussi». Se i proponenti concordano con questa riformulazione, il Governo

giustamente anticipato dal senatore Perduca, al cui ragionamento volevo ricollegarmi, ogni provvedimento che riguarda la Bielorussia dovrebbe essere occasione per ricordare

sull'efficacia dell'embargo, dell'isolamento economico come strumento di lotta contro chi nega i diritti umani.

onorevoli colleghi, qualche mese fa la Camera, che aveva già svolto un complesso lavoro di unificazione di testi presenti in materia,

(sulla spinta emotiva della gravità di fatti di cronaca che colpivano pesantemente la pubblica opinione) e quella di incidere in maniera significativa, anche alla luce dei disegni di legge presenti e giacenti in Senato, sul complesso della materia trattata. Quest'ultima fu la decisione che, dopo alcuni mesi di lavoro, può dirsi oggi giusta se presentiamo all'Aula un testo in larga parte condiviso e ricco di nuovi spunti e soluzioni. Un testo, direi, che sottende una filosofia, un pensiero, che non intende tradursi in un mero aumento delle pene, ma che con la previsione di nuove fattispecie, modulazioni e sfumature, e con 1'occhio attento ai mutamenti esponenziali della società e delle relazioni familiari intende porre l'accento sulla gravità crescente del fenomeno della pedofilia, della pedopornografia, della violenza sui minori e tra (sottolineo «tra») minori, e sui mezzi più efficaci per prevenirla e combatterla. Ringrazio subito, quindi, tutti quei colleghi che hanno inteso, appassionatamente (come potrebbe non essere così quando parliamo di bambini, di minori e di violenza!), contribuire ciascuno dal proprio e con il proprio punto di vista a migliorare il lavoro dei relatori. Il testo, senza tentennamenti ed anzi con maggiore assunzione di responsabilità rispetto a quello che la Camera ci aveva trasmesso, esamina il tema con verosimile completezza di prospettiva e punti di vista. Chiunque si affacci alla materia è tenuto a prendere tristemente confidenza con quegli articoli 600 e 609 del codice penale che, tra commi e lettere, rappresentano il campionario delle peggiori aberrazioni umane che sembrano trovare nei più recenti fatti di cronaca efficace quanto deprecabile vetrina. Ma qui il lavoro è stato più complesso perché si è tentato di incidere anche su problemi di competenza, di procedura, di applicazione di pena e di rito fino a pensare alla tutela del minore vittima nella fase processuale. Per una migliore comprensione del lavoro svolto dalle Commissioni in Senato e delle modifiche introdotte vorrei brevemente riassumere le caratteristiche salienti del testo che la Camera ci aveva trasmesso in relazione a quanto previsto dalla Convenzione, trascurando ogni aspetto che rilevi alla Commissione affari Sul piano del diritto sostanziale, vorrei ricordare l'inserimento nell'ordinamento dei reati di pedofilia culturale di cui all'articolo 414-*bis*, così come originariamente rubricato dalla Camera (sul quale, peraltro, tornerò nel prosieguo del mio intervento), da un lato, e di adescamento di minore anche tramite l'utilizzo della rete Internet (il cosiddetto *grooming*), di cui al nuovo articolo 609-*undecies*, dall'altro. A questo proposito, va sottolineato che il Senato, grazie ad una intelligente quanto caparbia intuizione del senatore Caruso, ha voluto sostituire la rubrica «pedofilia e pedopornografia culturale» con quella «istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia», a significare che in sé la pedofilia non può portare nulla di culturale e che non c'è nulla di culturale che la giustifichi. Tali nuove fattispecie di reato, cioè l'istigazione e l'adescamento, sono volte ad anticipare la soglia della punibilità, sanzionando tutti quei comportamenti che si verificano in momenti che precedono l'abuso. Si è voluto, in altri termini, prevedere nuove fattispecie in grado di combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia. Rilevanti modifiche sono state introdotte dalla Camera dei deputati anche in relazione al codice di rito. In particolare, vorrei segnalare che con la novella dell'articolo 282-*bis* si è intervenuti in materia di allontanamento dalla casa familiare attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l'applicazione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena. Vorrei altresì segnalare, da un lato, l'esclusione dell'applicazione del patteggiamento nel caso di prostituzione minorile e, dall'altro, le novelle apportate agli articoli 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*, in materia di incidente probatorio. Concludo la disamina delle principali modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, e sostanzialmente non riviste dalle Commissioni 2a e 3a del Senato, soffermandomi sull'articolo 9 che, così come per la violenza sessuale, anche per la pedofilia

di rilievo della Commissione affari esteri. Le restanti norme, incidendo sull'ordinamento giuridico nazionale, attengono - come già detto - all'ambito di competenza della Commissione giustizia. L'articolo 4 interviene sulle norme del codice penale relative ai delitti contro la libertà individuale e contro la libertà sessuale. In primo luogo si è intervenuti, modificando il testo approvato dalla Camera, sull'articolo 157 del codice penale, prevedendo un aumento dei termini di prescrizione per i delitti contro la libertà individuale, nonché per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo, ad eccezione dei casi di minore gravità. Significativa è l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. L'emendamento in oggetto, oltre ad avere modificato la rubrica dell'articolo come consegnataci dalla Camera, in modo ben più coerente con la logica sistematica del codice, ha inserito due nuovi commi con i quali, da un lato, si esclude la possibilità per il la possibilità per il reo di invocare a propria scusa ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume, e, dall'altro, si prevede un aumento di pena per i casi in cui il fatto sia compiuto avvalendosi del mezzo della stampa, anche telematica. Con un emendamento dei senatori Perduca e Poretti si è definitivamente sostituita la residuale definizione «pena di morte» con «ergastolo» nella rubrica dell'articolo 576. L'approvazione dell'emendamento Li Gotti ha arricchito il testo del disegno di legge con una significativa riscrittura dell'articolo 572 del codice penale in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Oltre ad un generale inasprimento del quadro sanzionatorio per la condotta tipica, si prevede un aumento della pena detentiva massima, da otto a nove anni, nel caso in cui dal fatto derivino lesioni personali gravi. Rispetto poi al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il disegno di legge in titolo interviene anche sul reato di cui all' articolo 583-*bis* (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). In particolare, con l'accoglimento di un di un emendamento Caruso sono state previste, quali sanzioni accessorie del reato suddetto, la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore, nonché l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura (per la verità già contemplate dall'articolo 602-*bis* del quale è stata contestualmente disposta l'abrogazione). A seguito dell'approvazione di tre distinte proposte emendative è stato anche incisivamente riscritto l'articolo 600-*bis*, in materia di prostituzione minorile. Oltre ad un inasprimento del quadro sanzionatorio è stata soppressa la circostanza attenuante rappresentata dalla minore età dell'autore del fatto, e ciò per significare che una violenza commessa da un minore su un minore non diminuisce certo il disvalore del fatto. Ancora, l'emendamento della relatrice 4.1000 è intervenuto sul reato di «pornografia minorile» di cui all'articolo 600-*ter*, introducendo nel testo la definizione di «pornografia minorile» e prevedendo pesanti sanzioni per coloro che assistono ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano stati coinvolti minori di diciotto anni. Nell'ambito della complessiva ridefinizione delle circostanze attenuanti e delle pene accessorie disposta dal disegno di legge così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, è stata reintrodotta la sanzione della chiusura degli esercizi commerciali e la revoca della licenza per le emittenti televisive la cui attività risulta finalizzata alla commissione di delitti contro la libertà individuale. Il già richiamato emendamento 4.21 Caruso è intervenuto incisivamente anche sull'articolo 602-*ter* recante le circostanze aggravanti, prevedendo in particolare aumenti di pena nei casi in cui i reati di violenza sessuale, di pornografia minorile, di turismo sessuale e di tratta siano commessi, fra l'altro, approfittando dello stato di necessità del minore, ovvero mediante la somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, ovvero nei confronti di minori in stato di infermità o minorazione. Di particolare rilievo sono poi le modifiche apportate al codice nei casi in cui si è previsto che per i di delitti contro la libertà individuale - quelli del 602-*quater* contro la libertà sessuale - 609-*sexies -* il colpevole non possa invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, qualora il fatto sia commesso in danno di un minore di anni diciotto e non già di un minore di anni sedici, come prevede invece la normativa vigente. Oltre ad interventi volti ad assicurare migliore sistematicità al testo, l'emendamento 4.2000 ha integrato l'articolo 609-*nonies,* prevedendo fra le pene accessorie da comminarsi ai colpevoli del reato di violenza sessuale, di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di atti sessuali con minorenne, di violenza sessuale di gruppo, di corruzione di minorenne l'applicazione di alcune misure di sicurezza personali, fra cui il divieto di svolgere lavori che prevedano contatti abituali con minori e l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Il disegno di legge all'articolo 5 reca modifiche anche al codice di rito, alcune delle quali legate all'esigenza di coordinare la disciplina processuale con la nuova normativa di diritto sostanziale. Al riguardo una significativa novità è stata introdotta grazie ad un emendamento del senatore Centaro, con il quale si è sottratta alle procure distrettuali la competenza sui procedimenti per i delitti di violenza sessuale, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di pornografia virtuale e di turismo sessuale. Il testo licenziato dalle Commissioni, poi, oltre a prevedere un aumento dei termini di durata massima delle indagini preliminari anche per i reati di prostituzione minorile e di pornografia minorile e l'estensione dell'istituto dell'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di persona minorenne nei procedimenti per i delitti in questione, ha introdotto, attraverso modifiche agli articoli 351, 362 e 391-*bis*, nel procedimento penale la figura del consulente tecnico esperto in psicologia e psichiatria infantile. L'articolo 6 del disegno di legge, recante modifiche alla legge n. 1423 del 1956 in materia di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dai minori non è stato oggetto di intervento da parte delle Commissioni riunite. Significative modifiche, invece, sono state apportate all'articolo 7 del disegno di legge, recante norme sull'ordinamento penitenziario. In particolare, con un emendamento dei senatori Li Gotti e Pedica, è stata prevista la possibilità per la magistratura di sorveglianza di valutare la positiva partecipazione a programmi di riabilitazione specifica per i detenuti e internati per i delitti di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di atti sessuali con minorenni nonché di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo a danno di minorenni. La relatrice, infine, con un emendamento ha promosso nella legge sull'ordinamento penitenziario di un nuovo articolo, il 13-*bis,* che prevede la facoltà per i condannati per reati sessuali in danno di minori di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. All'articolo 8 del disegno di legge in materia di confisca sono state introdotte modifiche sostanzialmente di coordinamento: infatti, la norma di cui all'originario comma 2 è stata inserita con analoga formulazione nell'articolo 600-*septies* del codice penale. Nessuna modifica, infine, è stata apportata al testo della Camera alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, recanti rispettivamente l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio e la clausola di invarianza finanziaria. Ecco, questo è il complesso lavoro che offriamo oggi all'attenzione dell'Aula quale punto finale di una riflessione a cui ciascuno di quanti hanno inteso attivamente partecipare è pervenuto attraverso la propria esperienza professionale, politica e di cittadino. Insomma, un testo che nella oggettiva difficoltà

secondo un'impostazione, all'interno di un quadro sistematico di norme, a cui l'Italia, diciamolo, certamente molto prima di Lanzarote, aveva inteso conformare la convivenza civile dei propri cittadini.

Si tratta del primo strumento internazionale con il quale gli abusi sessuali contro i minori diventano reati penali, compresi quelli che hanno luogo in casa o all'interno della famiglia, con l'uso della forza, con la coercizione o le minacce. La Convenzione include un preambolo e 50 articoli, divisi in 13 capitoli. Il preambolo richiama gli strumenti giuridici esistenti nel campo della protezione dei diritti dei minori, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991. Il Capitolo I individua l'oggetto della Convenzione e dunque la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, afferma il principio di non discriminazione e reca le definizioni. Per minore si intende ogni persona al di sotto dei 18 anni di età. Il Capitolo II riguarda le misure preventive. Le parti si impegnano a promuovere la consapevolezza dei diritti dei minori presso il personale che è a contatto con il mondo dell'infanzia, quali operatori del sistema educativo, delle forze dell'ordine, delle attività sportive. Le parti dovranno fare in modo che nei cicli di istruzione primaria e secondaria i minori ricevano le adeguate informazioni circa i rischi di sfruttamento sessuale e di abusi. Anche il pubblico dovrà essere informato e la Convenzione prevede che le parti incoraggino i minori, il settore privato, i media i media e la società civile a partecipare all'elaborazione delle politiche di prevenzione. Il Capitolo III prevede l'istituzione di organismi nazionali o locali per la promozione dei diritti del minore ed impone il loro coordinamento. Il Capitolo IV, in materia di protezione ed assistenza alle vittime, stabilisce l'istituzione di programmi e la creazione di strutture per fornire supporto ai minori vittime di abusi sessuali e ai loro parenti e affidatari. Viene prevista l'adozione di misure che consentano la segnalazione di sospetti e l'attivazione di linee telefoniche o Internet con operatori in grado di fornire assistenza. Il Capitolo V prevede l'adozione di programmi per persone processate o condannate per reati a carattere sessuale a danno dei minori, al fine di prevenire recidive. Il Capitolo VI elenca una serie di comportamenti che le parti si impegnano a considerare reati, relativamente agli abusi sessuali, la prostituzione e la pornografia infantile, la corruzione di bambini e l'adescamento a scopi sessuali, il favoreggiamento di tali reati. Il Capitolo VII stabilisce che indagini e procedimenti siano condotti nel rispetto dei diritti del minore. L'articolo 31 contiene un elenco di misure volte a proteggere le vittime e le loro famiglie nel corso delle indagini e dei procedimenti penali, tra cui la costante informazione sui diritti e sui servizi a disposizione e la possibilità di essere assistiti. È previsto che i reati siano perseguibili d'ufficio e che il procedimento continui anche nel caso in cui la vittima ritratti. Stanti le difficoltà di denunciare offese sessuali prima del compimento della maggiore età, la Convenzione prevede che i termini di prescrizione siano differiti per un periodo di tempo sufficiente a permettere l'avvio effettivo dei procedimenti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. Il Capitolo VIII dispone misure in materia di conservazione e registrazione dei dati a carattere personale. Il Capitolo IX stabilisce tra gli Stati membri una profonda cooperazione a carattere internazionale per prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali sui bambini, per proteggere le vittime e per perseguire i colpevoli. Il Capitolo X istituisce un meccanismo di monitoraggio affidato al Comitato delle parti, formato dai rappresentanti delle parti aderenti e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e di altri comitati intergovernativi. Il Capitolo XI disciplina i rapporti con altri strumenti internazionali. È stabilito che la Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalla Convenzione dell'ONU relativa ai diritti del minore, unitamente al suo protocollo opzionale concernente il traffico di minori e la prostituzione e la pornografia infantili, né da altri dispositivi ai quali le parti aderiscono. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea, e all'adesione degli altri Stati non membri. L'entrata in vigore è subordinata al deposito degli strumenti di ratifica di cinque Paesi, inclusi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa. La Convenzione non è ancora entrata in vigore poiché sinora solo Albania e Grecia hanno completato la procedura di ratifica. In conclusione, le Commissioni riunite propongono l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

È un documento di estrema importanza, e per rendersene conto basta porre mente a due passaggi del preambolo della Convenzione. «Lo sfruttamento sessuale dei bambini, in particolare sotto forma di pornografia infantile e di prostituzione, così come tutte le forme di abuso sessuale riferite ai bambini, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono gravemente in pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del bambino». recita come segue: «Lo sfruttamento e gli abusi sessuali riferiti ai bambini hanno raggiunto dimensioni inquietanti sia a livello nazionale che internazionale,

Sulla base di questo Preambolo, la Convenzione ha articolato diversi passaggi e sollecitazioni agli Stati nazionali, finalizzati al recepimento di queste indicazioni e quindi anche all'adeguamento interno della normativa già esistente. Il nostro Paese sicuramente non era in una posizione di scopertura su questo fronte: nel corso del tempo ci si era dati una normativa interna, ritenuta da più parti sufficiente. Tuttavia, bisognava ulteriormente intervenire, tant'è vero che nel corso dei lavori, sia alla Camera sia in Commissione al Senato, sono state approvate modifiche normative al nostro ordinamento interno, sì da rendere più puntuale la normativa nel rispetto del Preambolo che individua il bene che si intende tutelare. C'è un punto che è rimasto particolarmente scoperto, oltre ad altri, ed è quello per cui, nonostante nella stessa Convenzione ci si preoccupi di richiamare l'onere per tutte le parti di assicurare indagini e procedimenti efficaci per i reati stabiliti in conformità alla Convenzione il nostro Paese da anni, in questo settore di criminalità e di beni offesi come in altri settori, non riesce ancora ad ad approvare la normativa sulle squadre investigative sovranazionali, che sono le sole che consentono di superare le lentezze e la burocrazia dello strumento delle rogatorie. Specie in crimini come questi, ma anche per altri, è necessario che si arrivi ad individuare anche questo strumento d'indagine, che coinvolge di più Paesi interessati dalla medesima condotta criminosa. Purtroppo, da due anni si cerca di approvare tale normativa e il nostro Paese ancora non riesce a dotarsene, pur essendo i disegni di legge già stati esaminati nelle Commissioni. Pertanto, oggi approviamo il provvedimento in esame con modifiche all'ordinamento interno, sapendo che c'è qualcosa che ancora non abbiamo fatto, qualcosa che potevamo fare e che in questi due anni non si è trovato il tempo di fare. Non esiste la possibilità di aggredire questo crimine, che spesso viaggia anche attraverso forme di delinquenza transnazionale, se non ci si dota di uno strumento di indagine adeguato al tipo di crimine.

però chiamati a fare qualcosa di più e forse abbiamo perso l'occasione. Questo non vuol dire che non si possa ritornare sull'argomento e noi insisteremo, ovviamente, sugli emendamenti che avevamo presentato in Commissione e che abbiamo ripresentato in Aula, sperando che qualcosa di più si possa ancora fare e che qualcosa di ulteriore possa ancora fare l'altro ramo del Parlamento. Nel momento in cui, però, si va a ratificare una Convenzione, prevale la soddisfazione di essere riusciti, in tempi abbastanza brevi, ad approvare questo strumento, approvato approvato dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, cercando di fare il possibile rispetto a qualcosa che, così come illustreremo nel corso dei lavori di questa mattina, poteva ulteriormente essere fatto. In ogni modo, il lavoro svolto dalla Commissione e dai relatori è stato un lavoro encomiabile, del quale noi li ringraziamo. Speriamo di poter proseguire questo percorso positivo anche in quest'Aula.

Convenzione che definisce il minore come la persona che ha da zero a 18 anni. È un provvedimento importante, oserei dire importantissimo, perché, nel momento in cui si parla di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, non vi sono sostantivi e aggettivi che possano definire queste forme di violenza e questo orrore.

Con la ratifica di questa Convenzione noi andiamo ad integrare, a migliorare e, in alcuni casi, a confermare la legislazione che il nostro Paese fortunatamente

Questo è un segno di grande civiltà per il nostro continente, perché consente ai 47 Paesi del Consiglio d'Europa di uniformare la legislazione a livello sovranazionale, individuando sia un percorso comune dal punto di vista preventivo, sia le stesse fattispecie di reato, sia l'inasprimento della pena. ha anche una forte valenza di contrasto alle azioni poste in essere da realtà criminali organizzate a livello nazionale e internazionale, che proprio sulla pedopornografia fanno affari d'oro e che fino ad oggi in alcuni Paesi, rischiavano di restare impuniti. Si tratta, quindi, di una trattazione organica ed omogenea della materia, che consente di tutelare l'integrità femminile e maschile

stima che oggi l'incidenza di rapporti sessuali forzati e di altre forme di violenza che includono un contatto fisico si attesti, tra bambini e bambine sotto i 18 anni, rispettivamente a 73 milioni di casi per i bambini maschi

l'età media delle vittime si abbassa. La non denuncia è uno dei drammi di queste forme di violenza.

che cerca di sanare un dramma che si verifica all'interno della nostra società. C'è un punto della legge che risulta lacunoso. Mi riferisco all'articolo 10 invarianza finanziaria: forse serviva un po' più di coraggio da questo punto di vista. Non voglio entrare nel merito nel merito della punibilità delle diverse forme di violenza e quindi di reato, che speriamo non si vengano più a produrre grazie anche all'azione preventiva posta in essere. Desidero solo ricordare l'introduzione del delitto di adescamento di minorenni, il cosiddetto *grooming*, punito con la reclusione da uno a tre anni. La condotta del nuovo reato consiste nel compiere qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di 16 anni attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante Internet, o altre reti altre reti o mezzi di comunicazione. La fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico: il soggetto agente deve aver agito al fine di commettere delitti di sfruttamento sessuale di minore o delitto di violenza sessuale. Quest'ultima fattispecie rappresenta una novità assoluta, finalizzata a punire la condotta intenzionale di un adulto - questo è importantissimo - che attraverso Internet proponga a un minore di incontrarlo con l'intento di commettere uno dei reati che che sono stati prima ricordati. In questo modo si capisce anche la gravità di questo reato. Voglio ricordare, rileggendo per altri motivi un passo di una persona che probabilmente non ci si immaginerebbe di poter citare su questo argomento. Lo voglio citare perché è una delle persone che tutti abbiamo studiato: Goethe. Che cosa ci diceva questo grande letterato e poeta? Ci diceva che chi ha molto a che fare con i bambini scoprirà che nessuna azione esteriore resta senza influsso su di loro. È per questo che fortunatamente oggi noi approviamo questo disegno di legge. Poiché nessuna azione resta senza influsso sui minori, ci dobbiamo occupare anche di queste forme di reato che vengono esercitate. Il dilagare di questi abusi sessuali è quindi un fenomeno che va fermato, perché rischia di diventare un danno irreparabile. La nuova previsione ha una grande rilevanza, se si considera che le azioni volte ad adescare minori via Internet, sconosciute fino a poco tempo fa, stanno diventando un vero pericolo per i bambini e per gli adolescenti che attraverso la rete inconsapevolmente possono fare incontri drammatici e pericolosi. Se da un lato la rete certamente rappresenta una grande occasione di sviluppo e di relazioni per tutti noi e quindi anche per i minori (soprattutto per i minori, che hanno anche una maggiore facilità di interazione con questi strumenti informatici e con la rete), si rischiano però di consumare, attraverso questo strumento positivo, dei crimini inauditi. Purtroppo oggi la navigazione è diventata pericolosa e noi ci dobbiamo occupare anche di questo. È importante quindi agire dal punto di vista punitivo, ma soprattutto per quanto riguarda la prevenzione. Infatti, la Convenzione individua delle misure preventive, che vanno dallo *screening* al reclutamento e all'addestramento del personale, così da evitare l'insorgere di questi reati. Credo quindi, concludendo e consegnando il testo integrale dell'intervento, che possiamo dire di compiere un atto dovuto, necessario e utile perché la dignità del bambino, che è sopra i confini geografici e sopra le parti, non può e non deve più essere violata. Concludo con le parole di Kahlil Gibran, contenute in una delle sue opere più belle, anche spiritualmente più belle, le «Massime spirituali», là dove dice: «Dio mi liberi dalla saggezza che non piange, dalla filosofia che non ride, dall'orgoglio che non s'inchina davanti ad un bambino». Noi oggi con questo atto ci inchiniamo davanti ai bambini.

Questa forma di perversione sessuale ha ormai sviluppato nuove tipologie insidiose, quali la pedopornografia *on line* e il turismo pedofilo. A questo proposito, preannuncio che esamineremo un emendamento che abbiamo presentato, che

Questo provvedimento contiene risposte concrete in termini di prevenzione e di contrasto. Se mi consentite, è un provvedimento importante anche dal punto di vista simbolico perché introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico e nel codice penale la parola «pedofilia»,

dove si parla espressamente di condotte di istigazione a pratiche di pedofilia. Riteniamo che questo reato che introduciamo *ex novo* non sia un reato d'opinione, bensì un reato che punisce delle condotte particolarmente offensive e spregevoli.

1996. A distanza di oltre 14 anni, il Parlamento ha ritenuto opportuno e doveroso metter mano alle azioni di contrasto alla pedofilia, attraverso la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che è il primo strumento internazionale per combattere gli abusi sessuali sui minori e, dall'altro, intervenendo sull'ordinamento interno con modifiche molto importanti, sia di carattere penale che processuale. Ricordo tra di esse il raddoppio dei termini di prescrizione ed il tema delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; tema a noi particolarmente caro, sul quale interveniamo indicando espressamente che chi viene condannato per questo reato spregevole di mutilazione degli organi genitali femminili perde completamente la potestà genitoriale e viene interdetto perpetuamente da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e

è poi un articolo che riguarda le misure di sicurezza nei confronti di chi è stato condannato per delitti di pedofilia e a sfondo sessuale. Si dice che dopo l'esecuzione della pena per una durata di cinque anni - a tale riguardo proponiamo che venga approvato l'emendamento del senatore Caruso che propone una durata minima di cinque anni - si applichino misure di sicurezza nei confronti delle persone condannate, che sono anche socialmente pericolose. Queste misure di sicurezza sono: l'imposizione di restrizione dei movimenti della libera circolazione, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori, il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con i minori e l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. tratta di misure particolarmente importanti perché consentono di evitare la recidiva, che cioè queste persone socialmente pericolose possano commettere altri reati dello stesso tipo. C'è poi l'introduzione del reato di adescamento in rete, il cosiddetto *grooming*, attraverso una formulazione che va a colpire non solo la rete propriamente detta, ma qualsiasi altra forma, dagli SMS agli MMS, alle *chat*, ai *social network* e ai giochi *on line*. È quindi una formulazione che comprende qualsiasi condotta che possa essere punita a titolo di adescamento. Aggiungo il tema delle modifiche all'ordinamento penitenziario, sul quale siamo molto attenti perché in esse si parla espressamente di un programma terapeutico di recupero e sostegno del pedofilo; chiamatela come volete, per noi rimane la castrazione chimica, cioè quel programma terapeutico che serve ad evitare il rischio di recidiva.

Dunque, non più automatismi nella concessione degli innumerevoli benefici penitenziari di cui purtroppo è caratterizzato il nostro ordinamento penitenziario, ma la condizione che il pedofilo condannato per questo tipo di reati si sottoponga volontariamente a questa cura ed

sono in vacanza, pigiano pulsanti e sono semplicemente senatori *on* *demand*: non domandano, non fanno, non ambiscono, semplicemente poltriscono. questo tipo di affermazioni, fatte da colleghi che magari non si distinguono per un'attività frenetica in Commissione e in Aula, meriterebbero altro spazio che non quello offerto dai giornali.

Lavoriamo tutti i giorni su provvedimenti importanti: faccio parte della Commissione giustizia, che sta lavorando in questo momento alla riforma della professione forense e inoltre stiamo licenziando un provvedimento che, dopo 14 anni, interviene con azioni importantissime di prevenzione e contrasto della pedofilia, e ci sentiamo dire da colleghi che stiamo qui semplicemente a poltrire. Credo che questo sia un tema che debba essere affrontato dalla Presidenza, stigmatizzando questo modo di rovinare la reputazione di tutti noi che lavoriamo quotidianamente in quest'Aula e nelle Commissioni.

il tratto della violenza come pedofilia e abuso e il tratto della violenza come sfruttamento, cioè prostituzione, pedopornografia e turismo sessuale. sessuale. Dobbiamo quindi rilevare che la Convenzione di Lanzarote si caratterizza rispetto alla legislazione nazionale e a quella di altri Paesi europei nel

essa è importante anche perché definisce la violenza, sottolinea l'importanza della prevenzione e cura,

quanto sia stato importante prevedere la competenza della polizia postale, mentre in tanti altri campi di specializzazione ci sono molte carenze) e introduce i diritti della vittima e della tutela;

è una sproporzione di forze, così come abbiamo deciso di introdurre i reati di prostituzione minorile, di pedopornografia e di turismo sessuale di turismo sessuale quali nuove norme di riduzione in schiavitù, perché il minore non è in grado di opporsi alla prostituzione minorile, al turismo sessuale, alla pedopornografia dato l'enorme lo scarto tra un minore

È pertanto positivo tutto quello che abbiamo fatto dal punto di vista delle pene, dell'introduzione di nuovi reati, della concezione della vittima e dell'autore del reato. Ma

parte la pena, non avremo niente in mano per operare contro la recidiva e soprattutto per tutelare i minori e le persone che stanno loro accanto.

La violenza, in tutte le sue forme, da quella sessuale al maltrattamento, alla negligenza, all'abbandono affettivo, alla non cura, è negazione della personalità. Ora, è sempre orrendo trovarsi di fronte alla negazione che gli altri fanno di te, ma quando si è piccoli, quando si è bambini, ovviamente questa negazione pesa molto di più, perché il bambino non ha ancora sviluppato la sua personalità; è una personalità in formazione, non sa chi è e quindi non può far leva su ciò che è già stato per combattere la negazione della sua personalità. Dunque, nel momento in cui la personalità si nega, si procurano due danni gravissimi: la perdita dell'autostima, che è fondamentale per poter investire su se stessi; la disistima verso gli adulti che dovrebbero aiutare a vincere le paure. del 1998, sul turismo sessuale, abbiamo inserito il concetto di extraterritorialità: abbiamo detto che qualsiasi bambino del mondo, a prescindere dalla cittadinanza, deve essere protetto in ugual modo e qualsiasi reato compiuto da un cittadino italiano nei confronti dei bambini del mondo deve essere perseguito. Voi sapete che l'azione penale è limitata ai confini di uno Stato; nel momento in cui si supera questo limite, lo si fa per un valore superiore e qual è il valore superiore? È il concetto di persona, che va riconosciuto ad ogni bambino del mondo. Nella famiglia deve valere lo stesso principio: il bambino è un figlio, ma è soprattutto, dopo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1989, un cittadino, e quindi la comunità lo deve tutelare anche dalla violenza che viene perpetrata in famiglia. Il fatto che la violenza venga compiuta in famiglia non deve essere un'attenuante bensì un'aggravante. Come ha detto il professor Pinheiro, la violenza è un attacco alla personalità del minore e, se chi la compie ha un rapporto di affetto con lui, se ne indeboliscono le resistenze, inducendolo in un stato confusionale ancora più grande. L'umanità ha compiuto un grande progresso culturale e sociale riconoscendo la stagione dell'infanzia. Come famiglia, come scuola, come società, come legislatori siamo tenuti a restituire l'infanzia all'infanzia, a dare il tempo ai bambini di essere bambini e di sviluppare la loro personalità, proteggendone la formazione.

Il senatore Li Gotti ci ha pregato di accelerare l'intervento sulle squadre investigative sovranazionali: credo che questa sia l'intenzione della Commissione giustizia. Qualcuno ha sottolineato il ruolo e la qualità del lavoro svolto dalla polizia postale in questi anni, che sono straordinari; occupare di più, ad esempio proteggendo la figura dell'agente provocatore, che a volte è stato un po' bistrattato e non totalmente garantito.

il Governo si augura che venga approvata al più presto la ratifica della Convenzione, tenuto conto che con la Convenzione di Lanzarote vengono introdotti nell'ordinamento

Vi è però da dire che, dopo un testo predisposto dai relatori con il contribuito dell'intera Commissione, maggioranza ed opposizione, si è ritenuto di dare un adeguamento alle norme del nostro ordinamento, per rendere l'azione di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale sui minori molto più forte ed incisiva. Questa volontà dei relatori si è tradotta in un consenso generalizzato della Commissione, perché tutti i Gruppi maggioranza e opposizione - partivano dalla generale condivisione della necessità di una forte azione di contrasto allo sfruttamento e all'abuso sessuale sui minori. Tale condivisione generale è stata poi raccolta anche dal Governo che, nel dare parere favorevole ad una serie di emendamenti della maggioranza e dell'opposizione, ha tenuto conto di alcune linee fondamentali. Anche nel momento in cui il parere è stato contrario, tenuto conto, più che della non condivisione dell'aumento di pena - tanto per fare un esempio - della necessità di un coordinamento delle nuove norme rispetto al sistema ordinamentale di diritto penale. di diritto penale. Con l'ulteriore parere che i relatori si accingono a dare e al quale il Governo aderisce, per quanto concerne alcuni aspetti positivi di ulteriori miglioramenti che possono essere apportati in quest'Aula, si dà un nuovo testo, un nuovo ordinamento, molto compiuto, tale da tale da giustificare quel ritardo, che ovviamente si registrerà nell'approvazione della Convenzione, avendo il Senato scelto la strada di un intervento complessivo che ha modificato il testo approvato dalla Camera.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In ordine agli emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 5.100, 7.0.100 (limitatamente al comma 1-*bis*),

il primo emendamento che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea è il 4.100. Il sistema introdotto in questo disegno di legge prevede il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 del codice penale

su un reato gravissimo, quello dei maltrattamenti in famiglia, previsto dall'articolo 572 del codice penale, riteniamo che anche questa fattispecie di reato

a firma del senatore Caruso, che affronta il medesimo tema e che - a dire la verità - mi sembra meglio confezionato del mio. Si interviene

determinati crimini per i quali la condotta di istigazione a delinquere è particolarmente odiosa. mi trovo a dover parlare dell'emendamento 4.106, che affronta il medesimo problema con riferimento ad un'altra fattispecie di reato, ossia la possibilità di inserire i reati presi in considerazione per l'istigazione a delinquere anche per il reato di associazione a delinquere le due condotte devono essere correlate: l'istigazione a delinquere (articolo 414) e l'associazione a delinquere

determinate fattispecie di reato, non si vede poi perché poi nell'articolo 416 sull'associazione a delinquere non si debba prevedere il medesimo trattamento. Ecco la ragione dell'emendamento 4.106, che peraltro avevo formulato in coerenza con l'emendamento 4.102. Se invece è meglio formulato

riferimento ai maltrattamenti in famiglia. Una delle questioni che ha impegnato e continua ad impegnare la dottrina è

La dottrina si è interrogata sul fatto se ritenere l'evento morte determinato dai maltrattamenti un elemento costitutivo del reato di maltrattamenti oppure un evento esterno. Se si trattasse di un evento costitutivo,

di modificare l'articolo 572 del codice penale prevedendo che se i maltrattamenti, ossia quelle condotte che si prolungano nel tempo attraverso una serie di atti,

che determinano sofferenza, costrizione e poi la morte della vittima, devono essere condannati non con la pena sino a venti anni, ma con la pena prevista per l'omicidio aggravato,

di pedofilia e di pedopornografia)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-*bis,* 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater.*1, 600-*quinquies,* 609-*bis,* 609-*quater* e 609-*quinquies* è punito con la reclusione da tre a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma». Si tratta molto probabilmente di un emendamento, chiamiamolo, radicalmente libertario,

del controllo della libertà di espressione, pur tenendo naturalmente conto del contenuto di tale espressione. in un Paese come il nostro, dove esistono norme molto strette per quanto riguarda il comportamento su Internet, chiederei a relatore e Governo, quando esprimeranno il parere, che immagino sarà contrario relativamente a quest'emendamento, di voler chiarire che si tratta di responsabilità individuale della persona che utilizza Internet per commettere tale crimine. Infatti, grazie ad una legge che porta il nome del Presidente della Commissione antimafia, in Italia tale responsabilità penale viene ampliata anche all'Internet *provider.* Sappiamo che

acquisito probabilmente il parere contrario, se si potesse in qualche modo confermare che la responsabilità è individuale, non arrivando quindi a mettere in dubbio la neutralità dell'Internet *provider*, credo si aiuterebbe chi in futuro dovrà applicare queste nuove norme.

nuove tecnologie, il che credo debba sempre essere tenuto presente quando si va ad aumentare le pene, come si fa, purtroppo in molti casi, con l'approvazione di questo disegno di legge di

invariato il testo del primo comma del nuovo articolo 414-*bis* del codice penale rispetto alla formulazione contenuta nel testo base, cioè quello votato dalla Camera dei deputati. Il comma in questione continuerebbe quindi a contenere una parte che è tuttavia divenuta del tutto pleonastica, quando si dice: «con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione», alla luce del fatto che le Commissioni hanno poi approvato un emendamento che ha reso tali condotte come aggravante della condotta generale. Questo è il primo degli argomenti che gli emendamenti si propongono di affrontare. La seconda questione, invece, riguarda il minimo edittale, che è stato individuato nella maniera invariata da tre a cinque anni,

Per completezza, devo dire che questo problema si porrebbe anche rispetto alla fattispecie di istigazione ed apologia contemplate dal vigente articolo 414 del codice penale, ma non può esservi dubbio sul fatto che triplicare il minimo

nella maniera più sbrigativa, nel senso che propone, puramente e semplicemente, di sopprimere, al comma

capoverso. La proposta contenuta nell'emendamento 4.115 (che è più complesso) affronta un problema di coordinamento del testo, che è derivato dall'approvazione di altro emendamento, oggi contenuto nel testo base, che introduce la previsione generale dell'articolo

L'emendamento 4.118 è improntato a semplice tecnicalità. Si tratta di dare coordinamento alle disposizioni che, in questo momento, sono replicate nell'articolo 600*-septies* del codice penale e nel nuovo articolo 600*-septies*.2. L'emendamento propone l'integrazione di tutte le disposizioni in una norma che sembra essere più efficace. Non mi soffermo sul punto perché - ripeto - si tratta di una tecnicalità. Tuttavia, va richiamata l'attenzione dell'Aula sul fatto che il tema affrontato è quello della confisca dei beni, tema di cui abbiamo potuto constatare la centralità in questo e in altri provvedimenti esaminati dal Parlamento. L'emendamento 4.121 riguarda la circostanza attenuante. Anche in questo caso, la proposta emendativa ha finalità di coordinamento e, in particolare, è volta ad uniformare la formulazione dell'attenuante contenuta nel quarto comma dell'articolo 609-*quater*

Tale formulazione appare quella preferibile (o almeno a me è apparsa quella preferibile), alla luce di un disposto generale contenuto nell'articolo 65 del codice penale. Si tratta, onorevoli colleghi, di un problema apparentemente minore, che si potrebbe liquidare come eufonia complessiva del testo. un problema cui dobbiamo badare nel momento in cui mettiamo mano, con nuove norme, al codice penale, vale a dire ad un sistema complessivo il cui funzionamento è garantito dal fatto che tutte le norme rispondano a comuni denominatori. Analogamente, signor Presidente, l'emendamento 4.122 affronta il problema centrale delle misure di sicurezza. in particolare che le misure di sicurezza abbiano una durata minima di cinque anni. Il giudice non può applicare una misura di durata inferiore. La misura di sicurezza, proprio per la sua specialità, è stabilita dal legislatore. Il giudice ha un compito centrale, che non diminuisce né i suoi poteri né le sue competenze, che è quello di procedere all'esame della persona alla quale ha deciso di applicare la misura di sicurezza per verificare se sono venute meno le ragioni per cui

genera almeno due riflessioni. In primo luogo, viene ratificata una convenzione internazionale che in materia di minori chiude il suo ciclo di verifica nei singoli Stati un periodo di tre anni, per quanto riguarda il nostro Paese, dopo la sua firma. Non è un tempo breve, ma fa certamente dimenticare imbarazzanti ritardi che hanno caratterizzato in passato l'attività di ratifica e di recepimento nell'ordinamento interno di disposizioni importanti. Per tutte ricordo, proprio in argomento di minori, la Convenzione dell'Aja e la Convenzione di New York che, anche in materia di adozione internazionale e quindi in un contesto assai delicato, hanno visto la loro integrazione nel nostro

La seconda riflessione ha una portata sostanziale e concerne aspetti decisivi delle misure di contrasto previste, che hanno possibilità di diventare effettivamente efficaci, concrete e utilizzabili. Considerata la delicatezza intrinseca dell'argomento, l'odiosità evidente delle condotte oggetto di contrasto e di riflessione, l'allarme sociale che procurano, credo di dover dire che la senatrice Allegrini, relatrice in quest'Aula, il senatore Palmizio, chi ha svolto e chi svolgerà la medesima funzione alla Camera dei deputati, possano ragionevolmente ascriversi meriti reali per l'opera realizzata e per i risultati conseguiti. Non diversamente, il Governo, il senatore Caliendo per esso e gli altri suoi componenti al Ministero degli affari esteri e a quello della giustizia. Questa è una battuta conclusiva che a volte si ascolta nell'Aula del Senato. La ripeto volentieri, convintamente e senza piaggeria alcuna, in questa occasione, non senza nascondere la soddisfazione per un'attenzione e un lavoro che ho personalmente svolto a partire dalla XIII legislatura. Con la legge n. 296, votata nell'estate del 1998, furono accolte proposte che avevo avanzato e che furono fortemente innovative: il consumo di prostituzione minorile, disvalore ritenuto per la prima volta anche penalmente sensibile, per non dire del turismo sessuale e dello strumentario di contrasto che la relativa norma prevedeva, dall'agente provocatore al fatto commesso all'estero e quant'altro. Credo di dover concludere dicendo che, a volte, al nostro Paese viene contestata una certa latitanza rispetto ai gravi problemi. caso, ha ragione la senatrice Serafini quando prima rivendicava una posizione di avanguardia dell'Italia sia in Europa che nel mondo, con riferimento ad alcuni contrasti, come quelli qui previsti. Sono norme, quelle che cominciammo ad approvare nel 1998, che abbiamo perfezionato nel 2006,

importante e nuovo che oggi si registra nell'Aula del Senato è quello di una condivisione complessiva di idee, che nel passato non fu tale. Ricordo che nel 1998 le disposizioni sul turismo sessuale, nella contrarietà e perplessità dei colleghi senatori del Partito Democratico della Sinistra, passarono col voto decisivo del senatore Monticone, allora appartenente al Partito Popolare. Credo che anche lui ne sarà soddisfatto, alla luce di quello che oggi concludiamo.

già prevista dall'articolo 600-*quinquies* che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, della responsabilità penale di chi fruisce di questo spregevole fenomeno, di quella terribile piaga del turismo sessuale minorile. Chiedo al Governo e al relatore una valutazione, tenendo conto che, se stiamo andando verso la punizione del cliente della prostituzione adulta, mi pare il caso di valutare la punizione e la responsabilità penale anche del cliente della prostituzione minorile, soprattutto estera, in forza di turismo sessuale.

capisco l'intenzione del senatore Caruso, però «una durata di cinque anni» e «una durata non inferiore a cinque anni»

e sono contenta che finalmente una proposta di legge presentata dal Partito Democratico nella precedente legislatura e riproposta in questa sede trovi accoglimento in modo trasversale. *(Applausi dal Gruppo*

avevo anticipato una riformulazione in linea con l'emendamento 4.103, però essa riguarda due fattispecie: l'istigazione a delinquere e l'associazione a delinquere.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età, con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della potestà dei genitori o della tutela legale». Con questo disegno di legge abbiamo aumentato tutte le pene possibili e immaginabili; avremmo l'occasione di togliere un rimasuglio di un'era in cui esistevano i reati contro la morale. Credo che si andrebbe nella direzione della ratifica di oggi se riconoscessimo l'importanza della violazione di un diritto individuale piuttosto che della morale.

anche a seguito della Convenzione di Lanzarote, credo che il problema sia gestito in maniera diversa ed anche perché è stato depositato un disegno di legge che vuole, ancora una volta, cancellare l'incesto dal nostro codice penale. Credo si debba comunque prendere in considerazione il dibattito che non è teso soltanto alla modifica dei nostri codici ma anche, credo, ampiamente culturale.

è relativo agli attentati alla morale familiare commessi con il mezzo della stampa periodica. L'articolo citato recita: «Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti,

quasi. Passo dopo passo, credo si possa tornare a porre l'attenzione, come dovrebbe essere nelle democrazie liberali, sull'individuo o persona, comunque lo si voglia chiamare, piuttosto che sulla morale, ancorché morale familiare, che è stata più volte sollevata nel dibattito generale. Chiediamo quindi al Governo - se fosse possibile - di prendere in considerazione la riformulazione del parere contrario a questo emendamento e cancellare l'articolo 565 del codice penale, perché esso veramente, oltre ad essere anacronistico, non ha senso.

perché risolve un contrasto che non è solo dottrinario, ma anche della giurisprudenza. La Corte di cassazione, a volte ha seguito una via, a volte un'altra nel ritenere il reato di maltrattamenti, con le sue conseguenze, come reato autonomo oppure no. L'accertamento della preterintenzionalità e della premeditazione sappiamo essere un fatto complesso. Lo è meno nel caso in cui l'evento principale, in questo caso la morte, si colloca all'interno di un maltrattamento che è continuativo e sistematico e che, quindi, ha sempre il contenuto della premeditazione. Questo per dire che la pena superiore in questo caso, come proposto dal senatore Li Gotti, a me non sembra non corretta.

vorrei associarmi alla dichiarazione fatta dal senatore Caruso. la pena dell'ergastolo in questo caso quando, alla violazione sistematica della salute e della dignità della parte offesa, e quindi a maltrattamenti in famiglia, consegue la morte, può

Una delle ipotesi più gravi è quella in cui la morte della vittima è l'esito di una condotta vessatoria, punitiva, segregativa, fatta di torture e di sofferenze. Stiamo parlando di maltrattamenti che vengono distribuiti nel tempo, talmente gravi da provocare la morte della vittima. Questo è un omicidio qualificato da una condotta particolare.

all'ipotesi per cui, ritenuta la morte una circostanza aggravante dei maltrattamenti e concesse le attenuanti generiche equivalenti, si arrivava alla pena della reclusione sino a cinque anni. Erano le conseguenze di questo articolo scritto male! Nel momento in cui si riscrive il testo e si qualifica il reato per la gravità che esso contiene, riteniamo che la pena debba essere

**Il Senato non approva**.

dell'età della persona offesa non può valere quale scusante. La vicenda è ben nota anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale è intervenuta in questa materia e ha già dichiarato, in particolare con la sentenza n. 322 del 2007, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 609-*sexies*, che concerne l'ignoranza dell'età della persona offesa.

emergono gli stessi problemi. Innanzitutto, sussistono una questione di interpretazione ed un rischio di applicazione diversa da parte della magistratura, per quanto riguarda il significato di detta aggettivazione. In secondo luogo, riteniamo che il minore vada tutelato nella maniera più ampia possibile e, quindi, che sia sufficiente precisare precisare che si tratta soltanto di semplice ignoranza. Ricordo, infine, che è la stessa Corte costituzionale che pretende dall'agente eventualmente colpevole un particolare impegno nell'evitare la lesione

interpretazione, ogni volta che si è trattato di valutare l'ignoranza da parte del soggetto in materia penale - fosse ignoranza della legge o dell'età - la Corte ha sempre seguito lo stesso orientamento sulla inevitabilità.

«Conseguentemente» fino alla fine

ho fatto un rapido controllo, e quanto afferma il sottosegretario Caliendo è probabilmente corretto dal punto di vista sostanziale. Tuttavia, non vi è dubbio che gli articoli 207 e 208 del codice penale, che riguardano le misure di sicurezza in via generale, 217, 219, 221, 222, 223 e 228 - e probabilmente non ne ho trovati altri per mia mancanza - parlano di misura minima.

capitolando alle pretese inglesi di un mercato speculativo senza regole, per continuare a operare secondo gli interessi della City di Londra, dove hanno sede l'80 per cento dei fondi speculativi, mentre a Piazza affari il finanziere bretone Bolloré allunga i suoi tentacoli su Ligresti e Premafin, da quattro mesi (da 121 giorni) il Governo omette di nominare il presidente della CONSOB e di sostituire un commissario. Sarebbe come se a New York la SEC americana restasse per mesi senza presidente, in una fase di gravissima turbolenza dei mercati, perché la Casa Bianca ed il Congresso non trovano un compromesso accettabile sui candidati. In un articolo uscito oggi sul quotidiano «la Repubblica», intitolato «Mercati senza arbitro: quattro mesi di scandalo», il vice direttore Massimo Giannini dice testualmente: «Da tempo fioccano le candidature. Da Francesco Greco, il procuratore aggiunto gradito a Giulio Tremonti, ad Antonio Catricalà, presidente in transito all'Antitrust sponsorizzato da Gianni Letta». Nelle ultime settimane pareva che si fosse raggiunto un accordo sul nome del vice ministro Giuseppe Vegas che, secondo Giannini, non sarebbe «la migliore delle scelte possibili, visto che si tratta di un "tecnico" che proviene

da quattro mesi le beghe interne del Governo impediscano di trovare un accordo per nominare il sostituto di un presidente, che - naturalmente non tornerò

alcune settimane fa, sull'onda dell'indignazione per alcune dichiarazioni fatte da amministratori di un Comune piemontese e poi di una Provincia

«quel ragazzo disabile dovrebbe essere inserito in un diverso sistema socio-assistenziale di cura». In base alla seconda «i disabili ritardano lo svolgimento dei programmi scolastici. Più utile metterli in percorsi differenziati». l'Italia in cui vivo è un Paese civile, che sin dalla Costituzione tutela le persone diversamente abili. Nel dicembre 2007 Maria Clara Ori, non vedente, intervenne al Quirinale leggendo, grazie al sistema *braille*, gli articoli 2, 3 e 38, dedicati ai diritti dell'uomo, alla pari dignità sociale, al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione. Mi chiedo se da allora abbiamo fatto qualche passo avanti o dieci passi indietro. I segnali sono inquietanti. Chiedo ai Ministri competenti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno